comunicato che non c'è ancora traccia di alcuna relazione tecnica su tutti i recenti emendamenti del Governo e dei relatori, e dunque è assolutamente improbabile che la Commissione possa completare i lavori

sarebbe un'eccezione se si procedesse normalmente, secondo il decoro che dovrebbe caratterizzare i lavori parlamentari.

Grazie

forestali e del turismo e il Ministro della difesa. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Presidente, onorevole Ministro, il decreto sicurezza ha introdotto una novella dell'articolo 93, comma 1-*bis*, del codice della strada, che, salvo limitate eccezioni, prevede il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, con conseguenti pesanti sanzioni in caso di violazioni. La circolare n. 245 del 2019 del Ministero dell'interno, attuativa della suddetta norma, ha inspiegabilmente previsto per i cittadini europei che si possa tener conto anche della cosiddetta residenza normale. La definizione di «residenza normale», introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 118-*bis* del codice della strada, è mutuata in realtà dal diritto europeo e, in particolare, dall'articolo 12 della direttiva europea del 2006 sul rilascio delle patenti di guida allo scopo di facilitarne l'acquisto. Si tratta di una norma, per così dire, speciale, che nulla ha a che fare con la residenza anagrafica. Ad oggi, a causa della circolare del Ministero dell'interno e di tale utilizzo della definizione di residenza normale, le autorità competenti sanzionano i lavoratori stranieri, i cosiddetti stagionali - quelli, ad esempio, del settore alberghiero con contratti di lavoro in Italia di durata superiore a sessanta che, non essendo residenti in Italia, non dovrebbero essere ricompresi nel divieto e, quindi, nemmeno sanzionati. Per forza di cose, il divieto interessa in particolare le Regioni situate nelle zone di confine, tra cui il Südtirol, dove il rischio di incorrere in sanzioni è più diffuso e gli effetti negativi connessi all'applicazione della norma in maniera distorta sono maggiormente avvertiti dai cittadini e dai lavoratori, specialmente transfrontalieri. In occasione di un incontro informale con i tecnici del suo Ministero, avevamo ricevuto rassicurazioni in merito a una modifica della suddetta circolare, ma ancora nulla è stato fatto. Ministro, c'è da dire che la disciplina attualmente in vigore appare del tutto inadeguata, specie se applicata ad alcune situazioni che nulla hanno a che vedere

che escluda l'inspiegabile utilizzo della definizione di residenza normale. In generale, chiedo poi se non ritenga opportuno un intervento legislativo *ad hoc*, affinché siano definitivamente esclusi dal divieto anche tutti i soggetti e le categorie al momento attuale ingiustamente coinvolti e sanzionati.

non volevano punire gli autisti della Croce Bianca o i camerieri degli alberghi di confine - mi sembra evidente - ma avevano e hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale, al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali, nonché di evitare l'applicazione delle sanzioni del codice della strada (ciò è accaduto in migliaia di casi). Il divieto cui ho fatto riferimento è temperato da alcune eccezioni esplicitamente previste. Si tratta quindi di disposizioni importanti che, come riferito dagli stessi operatori di polizia, stanno già facendo registrare risultati positivi che sono certo nel tempo andranno a consolidarsi. In ogni caso, visto che nessuna norma nasce perfetta e se dei problemi arrivano dal territorio e da quest'Assemblea è nostro dovere affrontarli, gli uffici del Ministero hanno già fornito

quelli dimoranti nel territorio nazionale per almeno centottantacinque giorni all'anno per interessi professionali o personali) potrà essere superata in via amministrativa, precisando l'esclusione dei cittadini comunitari residenti all'estero dal campo d'applicazione del divieto di

infine assicurare che le criticità segnalate ed emerse nella fase di prima applicazione della normativa sono adeguatamente affrontate in modo da salvaguardare le poche, ma evidenti situazioni meritevoli di uno specifico trattamento derogatorio, fermo restando l'obiettivo di colpire le migliaia di condotte elusive degli obblighi di legge. In conclusione, senatrice Unterberger, la ringrazio e le assicuro che siamo assolutamente a disposizione per risolvere i residuali problemi segnalati, visto che adottiamo i decreti per semplificare la vita alle persone perbene e complicarla ai furbetti e alle persone permale.

disposizione che ha introdotto il principio di trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi all'origine dell'agricoltura. La costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione da molto tempo, sin dal luglio 2016, e fa parte addirittura del piano dell'ex ministro Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano,

L'esigenza di stabilire la Commissione nel Capoluogo della Capitanata è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile sia all'ingrosso sia all'origine continuano a non essere remunerativi per i nostri produttori,

Gli agricoltori denunciano ovviamente le politiche comunitarie che svantaggiano il grano siciliano, pugliese, lucano, molisano e abruzzese, costringendoli ad abbandonare i propri terreni, visto che i costi superano sempre più Pare dunque evidente l'opportunità di individuare a Foggia la sede di questa Commissione sul grano duro, senza alcun indugio verso le sperimentazioni, come pure è stato annunciato qualche giorno fa da alcuni esponenti del Governo. Tenuto conto che, nonostante la citata legge, il decreto attuativo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della precedente legislatura, questa commissione non è stata istituita, anche a causa di ostacoli frapposti da alcune organizzazioni, vi sono stati anche ricorsi presso i TAR e il Consiglio di Stato per annullare i listini della borsa merci di Foggia. Tale grave ritardo nell'attuazione della CUN sul grano duro a Foggia penalizza il processo di trasparenza e aggrava le condizioni delle imprese cerealicole del Mezzogiorno in particolare, senza consentire ai consumatori di avere anche orientamenti circa la qualità tossicologica dei prodotti. Il mondo agricolo e quello dei consumatori aspettano quindi, sotto questo profilo, un chiaro segnale da parte del Ministro per indire rapidamente la Commissione e soprattutto affidare all'Antitrust un'indagine che argini i fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza e verifichi il rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.

Signor Presidente, il sistema cerealicolo italiano riveste una grande importanza all'interno dell'intero settore agricolo nazionale, sia per l'estensione delle coltivazioni e per la formazione di una parte rilevante del fatturato, sia per il forte valore identitario che esprime. Proprio a tal fine, il Ministero è impegnato nel sostegno alla filiera grano-pasta e nel consolidamento dei rapporti tra i trasformatori e gli agricoltori, per garantire massima tutela ai consumatori.

per la formazione di un prezzo di riferimento valido a livello nazionale, che superi il sistema attuale di quotazione delle borse merci. Al fine di progredire nelle procedure e a fronte di una richiesta di filiera, il Ministero ha già tenuto il 14 marzo 2018 un tavolo tecnico e in data 21 marzo 2018 ha inviato ai partecipanti un questionario per stabilire alcune caratteristiche fondamentali della costituenda CUN sul grano duro, tra le quali la scelta della sede. tale tavolo tecnico sono state invitate le organizzazioni agricole e la rappresentanza della parte industriale di trasformazione, proprio per individuare congiuntamente un percorso utile di formazione della CUN, e alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione GranoSalus. Il Ministero ha ricevuto solo tre risposte al questionario, due delle quali contenenti la richiesta d'interrompere il percorso di formazione della CUN da parte delle rappresentanze della futura parte acquirente, nessuna risposta o indicazione invece, è stata inviata dall'associazione GranoSalus. Convinto dell'importanza dell'obiettivo di avere un prezzo indicativo più trasparente per chi produce fuori dai contratti di filiera, lo scorso dicembre, al tavolo della filiera grano pasta, ho ribadito la disponibilità alla creazione di una Commissione unica nazionale per il grano duro nell'ambito di una serie di azioni per il settore in tale direzione sta continuando il lavoro di dialogo tecnico con le parti. In merito al recepimento di una griglia di valutazione tossicologica della qualità del grano, anche a tutela dei consumatori, richiesta dall'interrogante, giova ricordare che quello immesso sul mercato deve rispettare per legge tutte le caratteristiche di sicurezza e salubrità previste dalla normativa europea e nazionale in materia. Per quanto concerne le indagini *antitrust,* ricordo che esse spettano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, in caso di pratiche sleali, provvede d'ufficio. Ribadisco comunque l'impegno del Ministero, per quanto di competenza, a evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi. Grazie Ministro, le cose non stanno esattamente in questi termini, perché è assurdo che l'agricoltura sia l'unico settore in cui a decidere i prezzi d'acquisto delle materie prime siano le controparti forti, ossia l'industria, la trasformazione e i commercianti. Ho depositato un disegno di legge per superare tale ostacolo, perché questa CUN non si farà mai, dal momento che alcune associazioni di categoria di parte industriale non vogliono un processo di trasparenza, che pure lo Stato italiano ha avviato, dopo anni di dure battaglie. È merito del MoVimento 5 Stelle aver introdotto, anche su nostra sollecitazione, questa norma, che stabilisce il principio di trasparenza. pertanto l'ostacolo è l'ostracismo da parte delle industrie, lo si può rimuovere anche accogliendo la proposta che ho presentato, che lei può trasformare in un decreto immediato: non è con i questionari, infatti, che riusciremo a convincere le industrie a ripartire equamente il valore aggiunto lungo la filiera.

cosa pensa davvero su questo fondamentale strumento di accordi bilaterali con un'importante Paese qual è il Canada. È una risposta politica quella che vogliamo, perché è una scelta che il Governo deve fare. Vogliamo sapere allora se siete d'accordo o meno con la ratifica, che ancora non è avvenuta,

prosieguo di questo accordo. Nelle scorse settimane abbiamo iniziato a incontrare alcune delle associazioni di categoria, quindi abbiamo cominciato a vedere insieme a loro come sta andando il CETA. Sappiamo benissimo che adesso ci sarà una revisione di medio termine e di conseguenza ci sarà anche la possibilità di interloquire con il Canada per vedere cosa si può modificare. In questo momento stiamo vedendo

l'*italian sounding* in Canada sia ancora permesso. Queste sono le due motivazioni per cui in questo momento esprimerei ancora parere negativo.

abbiamo una risposta fresca da cui partire nei ragionamenti. Mi permetto solo di fare una considerazione. Come lei ben sa, nei mesi scorsi è stata aggiunta all'elenco delle denominazioni protette anche quella del prosciutto di Carpegna, certificando in modo plastico che quanto molti avevano detto, cioè che questa tutela riguardava solo un numero ristretto di denominazioni d'origine, in realtà non è suffragato perché gli accordi dicono cose diverse. A mio

c'è da chiedersi quale altra strada ci sia per tutelare le denominazioni d'origine. Quindi, da questo punto di vista, credo che il chiarimento cui lei faceva riferimento sia sicuramente fondamentale per il CETA, ma credo anche per tutto il settore italiano votato all'*export*, che (proprio ieri abbiamo vissuto un momento di approfondimento su questo tema) ha nelle denominazioni di origine un patrimonio straordinario sia in termini economici, che in termini di ricaduta d'immagine sull'Italia.

un problema che si sta riproponendo dopo poco più di cinque mesi dall'approvazione, da parte di entrambi i rami del Parlamento, di una mozione con la quale chiedevamo al Governo di difendere il settore agroalimentare italiano nelle opportune sedi internazionali, in particolare nell'ambito dell'ONU e delle sue principali agenzie. Grazie al suo intervento e a quello delle nostre diplomazie, l'ONU è tornata sui suoi passi e ha dovuto ammettere che i nostri prodotti agroalimentari e le nostre eccellenze del *made in Italy* non sono così dannosi per la salute come dicevano. Oggi ci troviamo a dover discutere nuovamente di questo tema. Il 19 gennaio scorso è stata presentata ad Oslo la commissione Eat-Lancet su alimentazione, pianeta e salute, che si propone di trasformare il sistema globale della nutrizione. Tale commissione dispone di risorse economiche straordinarie, è collegata a una fondazione che gestisce oltre 30 miliardi di dollari e intende proporre stili alimentari lontani dal nostro modello della dieta mediterranea, stili basati solo su studi epidemiologici, senza avere alla base nessun fondamento clinico che ne certifichi l'efficacia e la salubrità. Questo modello risulta avere delle gravi carenze. I passaggi attraverso cui tale commissione vorrebbe realizzare i propri piani sono gravemente lesivi della libertà di scelta del consumatore, al punto da prevedere prima una guida delle scelte attraverso incentivi, poi una guida attraverso disincentivi (che vorrebbe dire tassare alcuni cibi), poi la restrizione tramite l'esclusione di alcuni prodotti dal mercato e infine addirittura l'eliminazione della scelta, sulla base del fatto che sarebbe lo Stato a indicare al consumatore quali sono i cibi salutari. Viene naturale pensare che dietro questo ennesimo attacco al *made in Italy* ci siano ben altri interessi e che sotto la copertura della salute umana si voglia invece colpire l'agricoltura e la filiera agroalimentare. Le chiediamo pertanto se e come intenda nuovamente intervenire per tutelare ancora una volta la filiera agroalimentare italiana nei confronti di un modello contrario alle abitudini e alle tradizioni alimentari. Sarebbe opportuno farlo anche attraverso campagne di informazione mirate, che consentano ai cittadini consumatori di valutare in modo obiettivo l'iniziativa di questa commissione, la cui propaganda purtroppo ha già attecchito presso diversi *media* all'estero e, alcuni, anche in Italia, al fine di evitare che i consumatori possano mettere in atto comportamenti alimentari nocivi per la loro salute. il Ministero ha sempre lavorato rispondendo nell'ottica della mozione che era stata approvata all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento.

che ha modificato la posizione originaria che la Commissione avrebbe presentato a nome di tutti gli Stati membri, ancora una volta contro l'agroalimentare italiano. L'azione della delegazione italiana è stata finalizzata a contrastare l'eventuale approvazione di nuove linee guida sull'etichettatura nutrizionale fronte pacco, che legittimano sistemi di etichettatura basati sulla classificazione cibi sani/cibi non sani, sistemi di etichettatura FOP a colori (il famoso semaforo), sistemi che attribuiscono un giudizio sintetico sulle qualità complessive dell'alimento (Nutri-score) e sistemi basati su indicatori di nocività. Per quanto riguarda nello specifico l'iniziativa Eat, una *startup no profit* dedicata alla trasformazione del sistema alimentare mondiale, quest'ultima è ormai nota per il rapporto della commissione Eat-Lancet «Diete salutari da sistema alimentare sostenibile», in cui viene affermata la necessità di modificare le abitudini alimentari mondiali verso regimi alimentari più dietetici, da un punto di vista non solo della salute pubblica ma, anche e soprattutto, di lotta al cambiamento climatico. Questo modello pone attenzione su un incremento a livello mondiale della produzione e del consumo dei cibi ritenuti salubri (frutta, verdura, cereali integrali, legumi e frutta secca) e una drastica riduzione, o totale eliminazione, del consumo dei cibi ritenuti dannosi (in particolare di carne rossa, ma anche di carne bianca, latticini, zuccheri e cereali raffinati). Sono previste diverse gradazioni di intervento pubblico per «cambiare il sistema alimentare globale», comprensive di misure più morbide e misure più drastiche, quali l'adozione di incentivi per alcune categorie di prodotti alimentari identificati come sani, e di disincentivi per le altre categorie merceologiche, fino alla totale eliminazione della libertà di scelta da parte del consumatore. Il rapporto della Commissione afferma che l'industria alimentare dovrebbe addirittura ritirare dal commercio i prodotti inappropriati e diversificare il proprio *business*. succitato ha suscitato forte preoccupazione, non solo da parte del Governo italiano, ma anche a livello imprenditoriale presso le organizzazioni agricole di categoria e di produttori agroalimentari. Le principali perplessità si incentrano sulla non adeguata fondatezza scientifica del rapporto e soprattutto sul carattere prescrittivo delle sue conclusioni e raccomandazioni.

alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata. L'Italia ha promosso, promuove e sempre promuoverà la dieta mediterranea, riconosciuta il 16 novembre del 2010 patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, per i suoi positivi effetti sulla salute e incoraggia i produttori a mantenere la qualità eccellente dei prodotti tradizionali italiani. La posizione concettuale espressa nel rapporto della Commissione Eat-Lancet potrebbe produrre effetti discriminatori soprattutto nei confronti di quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale (DOP e IGP), che sono obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori. di settembre 2019 a Parigi è prevista un'ulteriore iniziativa dei promotori della campagna Eat-Lancet nell'ambito di un *think tank* cui sono stati invitati diversi rappresentanti della Commissione europea. Non si mancherà in tale sede di intervenire per controbattere rispetto a questi tentativi di influire sui Governi e sulle competenti autorità regolatorie in varie parti del mondo per imporre una visione non suffragata da convincenti evidenze scientifiche e senz'altro controproducente per il mondo agricolo e i produttori di alimenti sani e di qualità come quelli italiani. Quanto sopra non esaurisce l'azione di tutela delle eccellenze agroalimentari nazionali, perché intendiamo mantenere alta l'attenzione in tutti i fori internazionali, FAO compresa, in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, con l'intento di imprimere incisività e determinazione al ruolo dell'Italia, salvaguardando il *made in Italy*.

sinceramente sia svilente, non solo per quest'Assemblea, non solo per i consumatori, ma soprattutto per i nostri agricoltori e per i nostri produttori, che si trovano già a combattere contro i continui cambiamenti climatici e contro la concorrenza sleale, *in primis* dei Paesi europei e poi dei Paesi extraeuropei. Colgo l'occasione anche per ricordare - e la ringraziamo - che le risorse messe a disposizione dell'agricoltura e del comparto agroalimentare da parte di questo Governo negli ultimi sei mesi ammontano ad oltre 1 miliardo di euro. Questo al fine di favorire le produzioni italiane, che sono di assoluta qualità.

Il ritorno alla terra è indubbiamente favorito da tutto questo. I problemi, naturalmente, non mancano, ma l'attenzione che lei porrà a tale argomento è fondamentale per le nostre produzioni, per la redditività dei nostri agricoltori e soprattutto per il consumatore finale. Prima i prodotti italiani, sempre. Grazie, signor Ministro.

Signor Presidente, signor Ministro, l'inclusione è il tema scelto quest'anno per la tradizionale parata militare ai Fori imperiali del 2 giugno. Un evento che di per sé è inclusivo, proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli italiani. Ma tra i compiti delle Forze armate ricordiamo: la difesa dello Stato, la sicurezza e la sovranità nazionale, la protezione dei confini della Patria, la costruzione e il mantenimento della pace nelle missioni internazionali, interventi in caso di calamità naturale, difesa collettiva in operazioni in ambienti complessi. Insomma, le Forze armate non sono né associazioni di volontariato, e non è loro compito istituzionale combattere l'emarginazione sociale, né scambiare fucili con borse di studio per la pace, come ha chiesto e proposto il presidente Conte. La parata del 2 giugno è, è, o dovrebbe essere, occasione per celebrare ed onorare l'impegno dei militari e rafforzare il senso dell'appartenenza nazionale. È proprio questa specificità delle Forze armate che andrebbe onorata e rispettata in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ricordando sempre, ogni giorno, che i militari sono servitori dello Stato e ambasciatori dell'Italia nelle missioni all'estero. L'aver dedicato la parata del 2 giugno al tema dell'inclusione ci sembra, signor Ministro, un'ipocrisia ideologica, un'alterazione politica e anche un mancato riconoscimento della vocazione principale delle Forze armate. Pur condividendo l'ottica che la strategia *dual use* non potrebbe essere diversa, riteniamo che

una sfilata, più dai colori arcobaleno che dai colori del Tricolore. Buona festa buonista, signor Ministro. *Peace and love*!

la risposta all'interrogazione oggi in discussione mi consente di chiarire con esattezza una questione oggetto di particolare interesse ed evidenza mediatica, nell'auspicio che tale intervento possa dissipare tutti i dubbi e non dia spazio a strumentalizzazioni e e interpretazioni di parte. La festa della Repubblica è la festa di tutti i cittadini e di tutti i militari che rappresentano la Repubblica e i valori di unità che essa sottende. Per tale motivo, come parte essenziale della Repubblica, i militari rappresentano l'incarnazione stessa dei principi e dei valori costitutivi dello Stato. Il concetto di inclusione è interno alla difesa. Inclusione vuol dire considerare come parte integrante della compagine difesa tutti i militari che hanno rischiato la vita per il servizio e che, ad esempio, si sono ammalati a seguito del loro impiego nei teatri operativi. Questi militari per tanto tempo non hanno trovato un riconoscimento formale e solo ora, finalmente, si sta facendo chiarezza sulla genesi delle patologie collegate all'esposizione ad agenti nocivi, con il preciso intento di ridurre al minimo, se non addirittura eliminare, ogni fattore di rischio per la salute dei militari impiegati. L'occasione di questa ricorrenza così speciale per la storia della Repubblica mi ha imposto di tenere tutti nella loro debita considerazione, affinché nessuno, nella difesa, debba rimanere indietro. Per tale motivo, nel corso della sfilata avremo con noi rappresentanti delle vittime del dovere e delle famiglie di coloro che sono caduti per il bene della Patria. Inclusione vuol dire che, per la prima volta, parteciperanno i civili della Difesa e per la prima volta la riserva selezionata. La diversità delle scelte e delle abilità è un patrimonio comune e rispettare l'autodeterminazione delle persone è necessario perché un Paese si mantenga vivo e competitivo, anche nella considerazione solidale per chi ha maggiormente pagato per il proprio impegno. Tali considerazioni e argomentazioni mi consentono di affermare che la dedica della parata della festa della Repubblica al tema dell'inclusione non possa costituire una sorta di una sorta di *deminutio* dei valori militari o un mancato riconoscimento della vocazione principale delle Forze armate. Anzi, è un ringraziamento dovuto a tutti coloro che hanno dato la vita e sacrificato parte importante di essa per servire la patria. È la festa degli eroi del Paese, anche di quelli che, ammalatisi per il servizio, sono transitati al ruolo civile. In tale ottica, il tema che ha ispirato l'organizzazione dei festeggiamenti per il 2 giugno mi pare del tutto coerente con la vocazione delle Forze armate ed in perfetta armonia con il dettato costituzionale.

colorata e la rende ancora più visibile. Io ho capito, signor Ministro, che lei si è vergognata di aver fatto capire che questa storia dell'inclusione fosse un attacco a chi ha altre visioni, per esempio sul tema dell'immigrazione, che fosse un attacco al suo presunto alleato Salvini. Adesso ha cercato di aggiustare tale

ha cercato per un anno di stare accanto al ministro Trenta e di spiegarle che il nemico non è Salvini o chissà chi altro ma che, purtroppo, il Ministro ha deciso di fare valutazioni diverse. Non lo dico io, lo dice il suo Sottosegretario. E stia tranquilla: Paglia e Luca Barisonzi, medaglie d'oro ferite in Afghanistan e in altre missioni, non hanno bisogno della sua inclusione, perché sono già nel cuore delle Forze armate e di tutti gli italiani, senza bisogno che lei dedichi loro il 2 giugno.

quasi che non siano tutti i militari, con il loro impegno, a difendere ogni giorno in armi la pace! Non sono certo amanti della guerra, i militari!

Signor Presidente, signor Ministro, a nome del gruppo di Forza Italia, desidero interrogarla sull'annosa e controversa questione che riguarda la dotazione d'arma relativa al programma di rinnovamento della nostra flotta aerea attraverso l'introduzione di caccia di nuova generazione, denominati F-35. Il Gruppo Forza Italia, come lei sicuramente sa, non ha mai nutrito alcun dubbio rispetto all'importanza strategica e industriale della partecipazione dell'Italia al programma degli F-35. Da parte del Governo però questa chiarezza non c'è, non c'è stata e non ci pare all'orizzonte. Sul tema degli F-35 infatti, come su molte altre questioni, si sta verificando una dinamica insolita: anche quando siete in due riuscite ad esprimere tre posizioni. infatti affermato che il programma relativo agli F-35 è irrinunciabile; Di Maio il 31 gennaio 2019 ha detto che assolutamente no, non si possono buttare via i soldi con gli F-35. Lei è stata più cauta, affermando che sta studiando e valutando (ed è da un anno che sta studiando). studiando). Dal momento che riteniamo che il programma sia utile e indispensabile sul piano industriale, sul piano dello sviluppo tecnologico, dell'occupazione e del miglioramento delle capacità di difesa dello spazio aereo italiano, le chiediamo tre cose:

se ritiene, in coerenza con i pareri tecnici che arrivano dall'Aeronautica militare e dal Ministero della difesa, che il programma di sviluppo e di produzione di caccia strategici di nuova generazione, denominati F-35, possa rappresentare, come dicono tutti, un'eccellenza sul piano militare e possa essere altresì un'opportunità per lo sviluppo tecnologico ed economico dell'industria italiana della difesa.

La scelta di partecipare al programma sin dalle sue fasi iniziali va letta nella duplice ottica di soddisfare le esigenze prioritarie di difesa nazionale e alleata attraverso un sistema d'arma dotato di elevata tecnologia in grado di svolgere funzioni multiruolo avanzate, che consenta alle Forze armate di mantenere un adeguato margine di superiorità tecnologica rispetto alle possibili minacce, nonché di assicurare all'industria nazionale l'accesso a tecnologie innovative e all'avanguardia con i correlati e adeguati ritorni industriali e la relativa crescita occupazionale. Va anche detto, tuttavia, che l'impegno finanziario per il programma F-35, così come era stato originariamente concepito, è di assoluta rilevanza nel quadro del *budget* per la difesa e per le finanze pubbliche, e pertanto deve essere attentamente analizzato in un'ottica di valutazione complessiva del rapporto costi-benefici. Pertanto, sin dal mio insediamento ho chiesto agli uffici tecnici competenti una valutazione approfondita del programma che tenga conto delle esigenze e delle capacità delle nostre Forze armate e dell'indotto occupazionale connesso, delle importanti ricadute imprenditoriali e di ulteriori variabili utili allo scopo di determinare una riflessione esaustiva sul *dossier*. Al momento, il Dicastero è autorizzato a procedere al completamento della prima fase del progetto, che vedrà la realizzazione e la consegna di 28 velivoli entro il 2022 (i velivoli sinora consegnati sono 13), i cui contratti sono stati completamente finanziati come da richieste del Joint Program Office. Le diverse articolazioni del Ministero della difesa coinvolte stanno, come dicevo, esaminando le conseguenze sul piano delle capacità e su quello industriale e occupazionale - dei possibili scenari derivanti dalla eventuale rimodulazione del profilo di acquisizione dei velivoli, ovvero del livello di partecipazione al programma. Ritengo sia assolutamente chiaro e condivisibile il fatto che qualsiasi valutazione politica che preceda un'approfondita valutazione tecnica rischi di apparire superficiale, approssimativa e incauta. Nel concludere, sento il dovere di puntualizzare che le decisioni sul futuro del programma non possono comunque - alla luce delle implicazioni di carattere strategico internazionale, industriali e occupazionali - essere demandate al solo Ministero della difesa. Reputo infatti necessaria al riguardo una valutazione corale che consenta all'Esecutivo di sostenere con coerenza una posizione rappresentativa di un impegno che nei fatti è di lungo termine.

Le ricordo, signor Ministro, che la Difesa non è un comparto secondario dello Stato, ma un bene comune dello Stato e dei cittadini e, come tale, non solo va preservato, ma deve essere anche oggetto di corretti e giusti investimenti.

ci portano perciò a temere che lei voglia, forse, far fare al programma F-35 la fine che ha fatto fare al programma dei droni della Piaggio Aerospace, un programma già in corso che è stato stoppato. Per carità, sono scelte ma non le condividiamo contrario - e lo voglio ribadire - che il programma F-35 a regime consentirà di assumere, di aumentare e migliorare le nostre capacità di difesa; consentirà all'Italia di progredire dal punto di vista tecnologico e sarà anche una grande risposta sul piano dell'evoluzione scientifica e dell'occupazione. Per tale ragione, a nome del Gruppo, esprimo insoddisfazione per la sua risposta, con l'auspicio che lei possa dedicare del tempo a tale questione e giungere finalmente alle ulteriori valutazioni necessarie per dare una risposta definitiva su questo programma, anche perché siamo diventati lo zimbello d'Europa.

con l'emergere dei primi episodi di militari italiani ammalatisi o deceduti al rientro dalle missioni in Bosnia Erzegovina e Kosovo, due Paesi dove la NATO, nel 1995 e nel 1999, aveva fatto uso di proiettili all'uranio impoverito. impoverito (DU); secondo i dati dell'Osservatorio militare ad oggi si contano nel nostro Paese almeno 4.000 reduci colpiti da patologie asbesto-correlate e 359 decessi; ad oggi, viene confermato dalla ricerca scientifica che questi proiettili sono pericolosi, sia per la radioattività emanata, sia per le nano-polveri tossiche che rilasciano nell'ambiente; continuano a verificarsi toccanti vicende umane legate a patologie contratte a causa di agenti patogeni, alle quali occorre dare costante attenzione e assicurare una doverosa ricerca della verità; da ultimo, nei giorni scorsi è apparsa, su alcuni organi di stampa, la notizia di un militare che si è tolto la vita, perché colpito da una patologia connessa all'esposizione all'uranio impoverito nel corso di alcune missioni all'estero, era stato costretto ad affrontare un lungo quanto penoso contenzioso con il Ministero della difesa; il Ministro in indirizzo ha avuto il coraggio

si chiede dunque di sapere quali siano tali provvedimenti concreti che il Ministro intende intraprendere per affrontare una problematica che tanta sofferenza ha provocato e continua a provocare nel personale militare, che ha messo a rischio la propria incolumità fisica per servire lo Stato e che lo Stato ha il dovere di tutelare. Signor Presidente, ringrazio la senatrice per questa domanda, che mi consente di illustrare la posizione della Difesa e la mia personale su un tema quanto mai delicato per la vita di ciascuno di noi: la tutela della salute. tema che assume ancor più rilievo per tutti quei lavoratori maggiormente esposti a rischi professionali e, tra questi, i militari. Individuare le cause delle patologie che abbiano colpito o possano colpire i militari è per noi una priorità assoluta e, nella stessa misura, ci sta a cuore manifestare

le conclusioni cui è pervenuta quella Commissione sono state considerate il punto da cui è partita l'attività del tavolo tecnico, per approfondire le criticità emerse in relazione all'esposizione a particolari fattori di rischio ambientale in ambito Difesa. Nei giorni scorsi il tavolo ha concluso la propria attività con la proposizione di una relazione finale e di un possibile testo normativo, che solo dopo aver ricevuto il parere di concordanza dei Dicasteri interessati inizierà il suo *iter* di approvazione. Le soluzioni individuate per rispondere alle richieste di coloro che si sono ammalati durante il servizio a causa dell'esposizione a sostanze nocive, incluso l'uranio, agiranno su diversi fronti. In primo luogo, si propone di invertire l'onere della prova, sollevando così il personale dal dover dimostrare di aver contratto la patologia per per effetto dell'esposizione a sostanze nocive durante il servizio. Sarà ora l'Amministrazione a dover dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la malattia derivi da altre cause, diverse da quelle di esposizione a fattori di rischio. Si propone inoltre l'adozione di procedure in grado di oggettivizzare il più possibile il procedimento presso le commissioni mediche territoriali o centrali, al fine di evitare il più possibile qualsivoglia disparità di trattamento tra casi similari. Si ritiene anche necessario intervenire su alcune criticità riconducibili a una pesante stratificazione normativa determinatasi negli anni, disegnando nuove modalità operative per snellire le procedure e ridurre i tempi di attesa per il personale interessato. La recente notizia riportata dai giornali sul ritrovamento di uranio nel midollo di un militare conferma - se mai ce ne fosse bisogno - che dobbiamo rispondere velocemente al dramma dei tanti militari e delle loro famiglie e rendere sempre più saldo il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione e il suo personale. Peraltro, con immensa soddisfazione ho appreso che di recente il Consiglio di Stato ha individuato la natura giuridica, i presupposti e l'ambito applicativo delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare (COM) e del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare (TUOM) che tutelano il personale civile e militare ammalatosi di alcune gravi patologie tumorali in quanto esposto a particolari fattori

la ringrazio per la risposta e soprattutto per le iniziative già intraprese e che sta intraprendendo, che dimostrano

esigenze che sono rimaste inevase e inascoltate per troppo tempo. È un cambio di direzione ancora più importante perché le sue rassicurazioni arrivano proprio alla vigilia della festa della Repubblica, ricorrenza che sarà dedicata, per sua espressa volontà, proprio alle vittime, ivi inclusi i militari italiani rientrati dai teatri operativi malati di cancro a causa dell'uranio impoverito e che meritano dallo Stato delle risposte. Noi, nonostante le malevole interpretazioni e le sceneggiate cui abbiamo dovuto assistere proprio in quest'Aula dagli oppositori di professione, siamo invece molto grati per le iniziative del Ministro e siamo veramente orgogliosi della sua scelta. Un disegno di legge per tutelare i diritti dei militari che si sono ammalati è un obiettivo condivisibile - credo - innovativo e ambizioso

anche in questa circostanza sarà pronto a sostenere e a tutelare il nostro personale militare.

a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.7 sul decreto-legge sblocca cantieri,

martedì 4 giugno, a partire dalle ore 9,30, con seduta senza orario di chiusura. Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario.

È nostro dovere ricordare in quest'Aula le 28 vittime di quel nefasto evento, i numerosi feriti, gli sfollati e i danni subiti dai territori delle Province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. Nel corso di questi anni, grazie allo spirito di abnegazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni, l'Emilia-Romagna è riuscita a risollevarsi in quelle zone, ripartendo con risultati economici ancora più positivi. Sono stati fatti grandi passi in avanti nel percorso della ricostruzione ed enorme è stato lo sforzo dispiegato in questi anni per ricostruire abitazioni, imprese, opere pubbliche e beni storici e artistici. Ricordo che, dal giorno dell'evento, non un giorno di scuola è stato perso e tutti gli alunni a settembre sono entrati a scuola, con continuità e tranquillità. Certamente Certamente ci sono ancora aspetti e questioni da risolvere. Dal gennaio 2019 lo stato di emergenza è cessato in 29 dei 59 Comuni colpiti dal sisma, mentre rimane ancora attivo lo stato di emergenza nei 30 Comuni più colpiti e danneggiati che formano il cratere ristretto.

positivi. Non ci siamo mai fermati di fronte a questo. Certo, c'è ancora molto da fare. Una ricostruzione così complessa richiederà ancora molto tempo per essere debitamente conclusa, ma la situazione di stallo politico, economico e sociale in cui versa questo Paese e le prospettive future sempre più confuse ed incerte evidentemente non aiutano nemmeno questo grande passo questo grande passo che è stato fatto con la ricostruzione. Il Partito Democratico, ovviamente, è pronto a continuare a lavorare in collaborazione per completare il processo di ricostruzione. Mi auguro che anche il Governo continuerà a darci una mano. La seduta è tolta